la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente, in relazione ai lavori della Commissione bilancio sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016. Domani mattina dalle ore 9,30 alle ore 11 saranno discusse le mozioni in materia di obesità, già all'ordine del giorno di oggi. Contestualmente, sono autorizzate a convocarsi la Commissione bilancio e la Commissione giustizia per l'esame rispettivamente della Nota di aggiornamento al DEF e del decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari. Alle ore 11 si svolgeranno le comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 20 e del 21 ottobre. Nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 16,30, sarà dunque esaminata la Nota di aggiornamento. Per entrambe le sedute di domani non è previsto l'orario di chiusura, fermo restando il contingentamento dei tempi. Nella seduta antimeridiana di giovedì saranno discusse la mozione sul contrasto al fenomeno del matrimonio forzato e ratifiche di accordi internazionali. Ferme restando le mozioni già calendarizzate per le sedute antimeridiane di martedì 18 e 25 ottobre, si aggiungono, per la seduta antimeridiana di martedì 8 novembre, mozioni sui tumori femminili e sul rinnovo dei contratti delle forze di polizia; per la seduta antimeridiana di martedì 15 novembre, mozioni sulle pensioni minime e sull'inquinamento olfattivo; nonché, per la seduta antimeridiana di martedì 22 novembre, mozioni sulla scuola. Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-legge sull'efficienza degli uffici giudiziari e di tre disegni di legge definiti dalla 7a Commissione permanente (Festival Verdi, Scienze geologiche, Casa Museo Gramsci). Nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre avrà luogo il *question time* con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nelle sedute comprese tra il 25 e il 27 ottobre saranno esaminati il collegato sul lavoro autonomo, nonché, ove conclusi dalle competenti Commissioni, i disegni di legge sui parchi e sulla protezione civile.

Signor Presidente, mi lasci innanzitutto dire che ormai ci troviamo di fronte a delle innovazioni e, di innovazione in innovazione, non so francamente dove andremo a finire.

ha deciso che era più opportuno farle soltanto alla Camera dei deputati. Le battute in questo caso potrebbero essere molte. Speriamo che domani pomeriggio non abbia ancora una volta

in Commissione giustizia dall'ottobre del 2013. Francamente, non comprendo il motivo per cui non si vuole portare

essendo arrivato solo oggi in Commissione. Se vogliamo dare un minimo di parvenza di effettiva partecipazione al processo

anzitutto ringraziare la maggioranza e i colleghi Capigruppo di maggioranza per averci ascoltato e aver inserito le nostre due mozioni sulla scuola. Come avevo detto anche in Conferenza dei Capigruppo,

Prima di tutto perché, nonostante i desideri del presidente Renzi, siamo ancora in un bicameralismo paritario, e di conseguenza riteniamo che se il presidente Renzi decide di andare alla Camera dei deputati per confrontarsi con i colleghi deputati sia giusto un passaggio anche al Senato. Siamo la stessa cosa: spiegatelo al presidente Renzi, che forse non l'ha ancora capito. Il secondo motivo per cui vogliamo stigmatizzare questa mancanza da parte del vostro Presidente del Consiglio, è il fatto che

Ci viene così in mente quel momento in cui, in quest'Aula del Senato, ci disse che sarebbe stato l'ultimo Presidente del Consiglio a chiederci la fiducia. Ce lo ha detto a suo tempo: quindi secondo lui - se sarà così secondo gli italiani, è una cosa diversa - non ci sarà più un Presidente del Consiglio che chiederà la fiducia al Senato. La nostra opinione, però, è che non ci sarà più un Presidente del Consiglio seduto lì,

ci sono due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica - ahimè, per lui - e molto probabilmente, grazie agli italiani, esse rimarranno anche oltre il suo mandato da Presidente del mi sforzerò di essere la più rapida possibile, perché le osservazioni politiche sull'innovazione che lei oggi

se c'era un'esigenza temporale e tempistica del Governo, le Camere, nella loro autonomia, avrebbero potuto tranquillamente

innovare oggi in questo modo una prassi e una procedura che finora ha regolato la vita delle due Assemblee del Parlamento. se questo è il frutto di un'alleanza che torna e ritorna, cioè di quello che un tempo veniva definito il patto del Nazareno, che come un fiume carsico si inabissa e poi riappare su una questione che appare appare semplice ma che in realtà rimette in discussione il ruolo della parità delle due Camere, se questo doveva essere, lo abbiamo visto oggi alla Conferenza dei Capigruppo. Per questo, pur comprendendo le ragioni anche della tempistica, che a volte è contro di noi e contro il lavoro che correttamente si tenta di svolgere (che lo faccia il Parlamento o l'Esecutivo), il Governo

perché questa innovazione doveva partire esattamente dal Senato e domani? E se invece, come io ho adombrato, tutto questo nascondeva probabilmente qualche altra preoccupazione, qualche qualche altro problema su tre grandi questioni che vengo rapidamente ad elencare? Mi riferisco innanzitutto al dover affrontare tra stasera e domani il delicatissimo tema del DEF, sul quale questo Governo zoppica da tutte le parti. Il secondo è che un calendario doveva essere completamente svuotato dei due grandi temi che, oltre al DEF, angosciano la vita di questo Governo, sulla concorrenza, che evidentemente deve sparire dai radar di quest'Assemblea parlamentare, perché il Governo non è in grado di esprimere coerentemente

Questo è un tema quanto mai rilevante, ma ce n'è uno ancora più angosciante per il Presidente del Consiglio, che è la è la prescrizione e la grande questione che si è aperta con la magistratura nel confronto serrato su questo tema.

problemi degli italiani (che ne hanno tre o quattro di grandi problemi), tra cui innanzitutto la loro vita economica e la loro vita all'interno di una crisi drammatica che evidentemente non interessa né al Governo né al Parlamento, altrimenti qualcuno di questi temi, in una fase come quella attuale, avremmo potuto trattarlo. Ecco perché io ribadisco la nostra totale contrarietà a questo calendario di perditempo. Questo è un calendario per perdere il tempo e per coprire il Governo e le sue incapacità. Ribadisco ancorché la mia proposta di poter calendarizzare quanto prima la discussione di ben 13 disegni di legge sull'istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario italiano perché, come ho già detto, signor Presidente, da qui a qualche settimana il Paese scoprirà, con grande stupore di questo Parlamento,

avuto cognizione di cosa sia accaduto negli ultimi due anni nel nostro sistema bancario, dentro le nostre banche. Infatti, caro presidente Marino, giace e e dorme un sonno tranquillo un'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano: l'unico modo che avevate per rinviare la trattazione di un tema delicato e importante,

ci propone e vuole farci sorbire. Chiaramente, abbiamo evidenza da ogni punto di vista che tutta la discussione e quanto avverrà nelle prossime settimane sarà solo finalizzato alla falsa propaganda che il Presidente del Consiglio sta facendo per convincere gli italiani della bontà e della capacità del suo Governo. Se infatti il suo Governo fosse serio, signor continuerebbe il lavoro già iniziato qui in Aula in merito alla riforma del processo penale, di cui le chiedo che venga ricalendarizzato subito, alla ripresa

se non fosse una priorità. Poi ci troviamo il Presidente del Consiglio dei ministri che va in televisione, un giorno sì e l'altro pure, a dire che questo Paese ha bisogno di riforme per diventare un Paese certo, a partire da quelli che sono i tempi della giustizia. E poi il processo penale viene parcheggiato lì nell'angolo. Forse perché deve assumersi delle responsabilità e dire dei sì o dei no, che in questo caso possono non corrispondere a quella che lui vorrebbe fosse l'opinione degli italiani in merito al sì o al no, perché prevarrà il no. Presidente, aggiungo subito un'altra buona ragione per la quale ci saremmo aspettati questo calendario e non un calendario dei lavori serio. In Commissione finanze, infatti, giace da tempo una sfilza di disegni di legge in merito alla revisione dei rapporti del sistema bancario, per la separazione del sistema bancario speculativo da quello commerciale. Vede, signor Presidente, è il cosiddetto è il cosiddetto sistema che sta facendo andare a male tutto il sistema bancario: la speculazione. Su questo io le chiedo che vengano portati in Assemblea, subito, tutti i disegni di legge che riguardano la separazione bancaria, perché è ora che questo provvedimento sia affrontato e che il Presidente del Consiglio dei ministri venga qui dentro a giustificare le ragioni per le quali, quando gli interessa, le banche non sono un problema e si fanno perciò i decreti-legge di notte a Palazzo Chigi, e, quando invece interessano ai cittadini, i provvedimenti vengono lasciati giacere chiusi negli armadi. Sono i suoi scheletri nell'armadio riguardo alle banche e ai suoi rapporti torbidi con il sistema finanziario che non vuole affrontare qui in Aula e, quindi, nega ai cittadini il diritto di vedere protetti i propri

proprio il Presidente del Consiglio e la maggioranza che lo sostiene applaudivano nei giorni del terremoto, quando erano lì a rischiare la vita, come avevano già fatto precedentemente e fanno tutti i giorni, per salvare i nostri concittadini in difficoltà, ma che si dimenticano bene di considerare quando si tratta di dare certezze a coloro che oggi sono discontinui e non sono stabilizzati, e i sotto organici: ci sono più di 50.000 posti vacanti, nel nostro Paese, riguardo ai Vigili del fuoco. Oggi ci sono Vigili del fuoco che attendono di essere stabilizzati e posti vacanti. Qual è la ragione per la quale non viene data risposta e non vengono considerate queste come priorità? Forse perché non sono abbastanza per poter soddisfare il consenso elettorale del Presidente del Consiglio? Forse perché sono stati presi in giro più volte, con ammiccamenti e strizzate d'occhio che poi non si sono concluse, e adesso il Presidente del Consiglio ha vergogna ad affrontare il tema qui in Aula? Sono molto perplesso, ma non sono per niente stupito di come si stanno evolvendo i lavori, perché quella figura di cartone che domani non siederà qui in Aula, andrà invece in giro per il Paese a dire che tutto sta funzionando per il meglio. Nel mese di agosto la FIAT ha fatturato il 40 per cento in più di autoveicoli senza accorgersi che la gente non ha più i soldi per comprare gli autoveicoli perché, come si trova scritto su qualche muro, ormai la gente è costretta ad andare a lavorare per guadagnare i soldi per comprare l'automobile per andare a lavorare, per avere i soldi per comprare l'automobile per andare a lavorare: si crea un circuito vizioso che è lo stesso per cui, Presidente, alla fine al Paese viene nascosto che 107.000 giovani cittadini italiani sono dovuti emigrare all'estero per trovare lavoro, mentre il Governo sta importando 150.000-160.000 clandestini ogni anno, perché ormai fanno fatturato e garantiscono quello quello pseudoconsenso elettorale che vuole garantire al Presidente del Consiglio dei Ministri, non eletto e nominato da Napolitano, di poter contare sul consenso elettorale. Chiediamo la rapida calendarizzazione di questi provvedimenti e da qui si vedrà se interesse del Governo è il bene dei cittadini o semplicemente cercare consenso elettorale spicciolo con delle marchette.

l'inconsistenza di una maggioranza che non c'è e un reale problema politico. Credo che questo vada ulteriormente stigmatizzato e vada sottolineato, perché i cittadini devono sapere che i provvedimenti importanti, che cambiano la loro vita, neanche vengono presi in considerazione. Come sempre, ritengo sia estremamente importante portare in quest'Aula

quando dice che questo calendario dei lavori è stato predisposto per perdere tempo. No, non è così.

È un calendario che prevede la trattazione del decreto-legge n. 168 del 2016. Ella, signor Presidente, ha ricordato che i decreti-legge hanno una priorità

il decreto-legge è del 31 agosto 2016 e la Camera lo ha approvato e trasmesso al Senato in data 6 ottobre 2016, vale a dire dopo giorni. In questi trentasei giorni la Camera dei deputati ha apportato una serie di modificazioni a tutta quella parte che va a regolamentare il ricorso per Cassazione. Presidente, in Commissione giustizia non abbiamo neanche iniziato l'esame del decreto-legge, tant'è che la Commissione affari costituzionali,

Noi non abbiamo ancora il parere della Commissione affari costituzionali, parere particolarmente importante se, *prima facie*, almeno all'occhio di ciascun operatore del diritto, appaiono profili di dubbia costituzionalità. Ebbene, a noi non restano che pochi giorni non restano che pochi giorni per esaminare un provvedimento così complesso che va ad intervenire sull'articolo 375 e su altri del codice di procedura civile, in particolare sul tema del ricorso per Cassazione.

intervento per fare in modo che il decreto decada. Peraltro, non sarebbe onesto da parte mia, se si considera che non l'ho ancora approfondito approfondito e studiato; non è detto che io non lo condivida, quindi per quale ragione dovrei con un'attività ostruzionistica farlo decadere?

Non c'è dato il tempo di apportare altre modifiche, questo è chiaro, ma se proprio dobbiamo votare questo testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, senza avere la possibilità di eventualmente in qualche parte, perlomeno ci sia dato il tempo di convincerci della bontà del provvedimento! Ci diano il tempo di leggere il parere delle altre Commissioni impegnate e interessate.

Concludo, con una premessa monca, resa tale dalla sua Presidenza: la nostra proposta è di spostare

facoltà, senatore Mauro. Richiamo alla brevità nell'indicazione delle modifiche

e che è reso sempre più esplicito. Tuttavia, devo dire anche che concordo con la saggezza dei Capigruppo di maggioranza e anche di coloro che, nell'opposizione, hanno voluto convenire nel merito, di consentire al Presidente del Consiglio di non venire in Senato. Perché lo dico? Perché il bicameralismo paritario ha un effetto sconsiderato sul Presidente del Consiglio. Infatti, essendo costretto ad ascoltare precedentemente l'opinione della Camera e poi quella del Senato, quando va a Bruxelles cosa fa? Quando si riunisce il Consiglio, dice sempre: «Sì, sì, sì», soprattutto alla signora Merkel; fuori dal Consiglio, prende coraggiosamente la parola, perché forse ha ascoltato l'altro ramo del Parlamento, e parla contro Hollande e contro la Merkel. Credo quindi che, non essendo più obbligato a parlare con i due rami del Parlamento, finalmente prenderà posizione una sola volta.

LN-Aut e CoR).* Come non ci hai rappresentato quando hai fatto un fragoroso fracasso, termine spagnolo che significa disastro,

il Daspo per i politici corrotti, quello che non permetterebbe più di riciclarvi anche nelle partecipate.

che il Senato della Repubblica non si occupi del tema delle banche. Vorrei quindi che non risultasse soltanto la voce di coloro che dicono che è così, con un intento parziale e finalizzato

situazione che viene rappresentata dovesse essere affrontata in questa Assemblea, ci sarebbero gli strumenti a disposizione dei colleghi e dei membri della 6a

qualora fosse venuta in Commissione. Lei ha voluto coinvolgere l'Assemblea e mi sembrava giusto specificare in questa sede che, oltretutto con la collaborazione di tutti i Gruppi presenti, c'è un livello di attenzione che penso sia in linea con lo stile

una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo cui è stata legata. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. L'emergenza continua: altre tre donne sono state vittime di femminicidio in questi ultimi giorni. Il 5 ottobre a Riccione, in provincia di Rimini, Olga Matei, di quarantasei anni, è stata strangolata da un uomo con il quale aveva da poco tempo iniziato una relazione, Il giorno dopo a Ghemme, in Provincia di Novara, è stata accoltellata dal convivente Olga Shugai, di Ieri, infine, a Torino un'altra donna, Santina Lodi di settant'anni, è stata trovata morta nella sua abitazione: il marito ha confessato di averla uccisa a calci e pugni (con inaudita violenza, hanno riscontrato i Carabinieri). Salgono così a 17 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata il 30 giugno scorso. Molto spesso il femminicidio, voglio ricordarlo, viene descritto dai *mass media* come un gesto estremo, frutto della gelosia, della paura, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. Una descrizione che spesso quindi addossa anche alla donna, la vittima, una parte di responsabilità, in quanto colpevole di aver suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Si tratta di cieca violenza e volontà di dominio da parte di chi considera la donna non come persona, ma come proprietà. Per questo, penso che l'impegno più grande debba essere sul versante culturale, per educare al rispetto e alla parità fra uomo e donna; un impegno che deve mobilitare tutti, donne e uomini, istituzioni e tutti i settori della società. Per questo, considero molto importante e preziosa l'attività delle associazioni che in tanti centri del nostro Paese si battono per contrastare la violenza sulle donne. Per questo, considero fondamentale che si dia attuazione alla previsione dell'educazione alla parità di genere, prevista dal comma 16, dell'articolo 1, della legge chiamata buona scuola. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, è è stato riconosciuta la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Il nostro Parlamento ha quindi riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale, che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra donne e uomini. Per questo la si può e la si deve prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Occorre ora, però, monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Per questo, riproponiamo con convinzione il nostro appello, un appello alla Ministra con la delega per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e soprattutto dia piena ed accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello a tutto il Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno. Non possiamo più accettare questa mattanza. Signor Presidente, colleghi, vi parlo di una vittoria in una battaglia di giustizia fiscale. A febbraio 2016 una sentenza della Corte di cassazione ha messo finalmente la parola «fine» a una storia che dura ormai da molti anni, dicendo una volta per tutte che le piattaforme petrolifere a largo delle coste siciliane devono pagare l'IMU come qualsiasi altra attività produttiva. L'azione della magistratura ha seguito il grande lavoro di accertamento della Guardia di finanza in questi anni, che ha messo in luce un enorme fenomeno di elusione fiscale (ICI e IMU) da parte delle compagnie petrolifere. Sulla questione noi del Movimento 5 Stelle avevamo già presentato una interrogazione per chiedere al Governo chiarimenti in merito, ma pochi giorni fa è arrivata la Suprema corte, che si è pronunciata altre due volte, dando ragione ad altri Comuni e spazzando via ogni perplessità sulla questione, contribuendo quindi a scrivere una nuova pagina sul diritto delle comunità locali.

enorme. Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo esprimere soddisfazione per il prezioso lavoro svolto dalla Guardia di finanza, soprattutto dal nucleo operativo di Scicli, invitando l'intero corpo a non mollare e a proseguire in questa azione di accertamento, che probabilmente avrà altre fasi.

Ribadiamo il nostro impegno per vigilare affinché il Governo non cambi ancora le carte in tavola e non faccia l'ennesimo favore ai petrolieri, come sta già cercando di fare: le piattaforme, oggi e sempre, dovranno pagare esattamente come qualsiasi altro imprenditore, piccolo artigiano o agricoltore, che ogni anno paga l'IMU al proprio Comune. Nessun privilegio ingiustificato per i petrolieri.